nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signor Presidente, la nostra mozione può sembrare sfasata rispetto ai tempi in cui viene in discussione discussione e fin troppo incardinata sul calendario di politica internazionale di qualche mese fa. Del resto, queste sono le fantasie dei calendari parlamentari. però che di queste fantasie bisogna anche cogliere le opportunità. La nostra mozione risale a quest'inverno, al viaggio in Israele che fece il Presidente del Consiglio, accompagnato da altri Ministri, nasce dalle reazioni politico-diplomatiche a dir poco "atomiche" che quel viaggio suscitò nei nostri rapporti con la Repubblica iraniana

un rapporto non per questo dettato da inimicizie e ostilità pregiudiziali nei confronti della Repubblica iraniana. Oggi ci troviamo in una fase rende ancora più attuali quelle prospettive che allora sembravano dettate dalla cronaca. Spero che ciò consenta al Senato, grazie anche al contributo delle mozioni presentate successivamente alla nostra e all'aggiornamento ed affinamento della nostra, di incidere pienamente, tra l'altro in una giornata in cui la questione Israele-Medio Oriente è al centro di un'importante discussione

l'Iran, nella nostra mozione ci si preoccupa però di non abbassare di un centimetro la guardia rispetto alla cosiddetta lista nera: *black list* è il termine utilizzato dalla politica e dalla diplomazia degli Stati Uniti. Il Governo statunitense ha definito da tempo la Guardia rivoluzionaria iraniana "forza proliferatrice di armi di distruzione di massa" e "sostenitore del terrorismo" il suo braccio operativo all'estero.

che nella seconda settimana di settembre l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ospita un discorso del presidente Ahmadinejad da cui emerge il

ha voluto sin dal suo insediamento riprendere le fila di quella che dal 2001 al 2006 era stata una costante, rapporti di amicizia e massima intransigenza sul diritto all'esistenza dello Stato di Israele, senza quei cedimenti che nella storia d'Italia si sono affacciati, una volta da parte dell'Ente nazionale idrocarburi, una volta con certe complicità con con certe complicità con gli eccessi di antisionismo delle Nazioni Unite. Da questo punto di vista, noi ci troviamo nelle settimane nelle quali c'è un appuntamento di politica internazionale

istituita fin dal 1948, è da qualche mese caratterizzata dalla presenza di un alto commissario del nostro Paese, che era già stato a lungo vice commissario. il presidente Dini e altri colleghi ne abbiamo ascoltato le dichiarazioni programmatiche qualche settimana fa in Commissione esteri. Nel descrivere storia e funzione di questa UNRWA, ovviamente senza esprimerlo in una mozione, perché è estraneo agli usi del Senato, nutriamo nessuno spirito di polemica nei confronti di Filippo Grandi che, come suo legittimo diritto, ha interloquito in un'intervista alla stampa polemizzando con l'opportunità della mozione Gasparri, allora l'unica esistente. quanto Filippo Grandi ha riferito alla Commissione affari esteri, la riduzione dei finanziamenti occidentali e le restrizioni imposte da Israele alle importazioni per Gaza

Noi prendiamo atto di ciò, almeno come dichiarazione di buona volontà del funzionario italiano. Abbiamo però avuto una sensazione malinconica, perché proprio da un funzionario italiano ci aspettavamo un richiamo

delle pur meritorie affermazioni che facemmo il collega Marcenaro ed io in quest'Aula a suo tempo e che mi paiono riprese nella mozione dei colleghi della sinistra. Anche se, a proposito della liberazione di Gilad Shalit, nelle mozioni della sinistra opportunamente si fa riferimento a uno scambio

da parte del dottor Filippo Grandi, tanta attenzione a esplicitare l'inopportunità della mozione Gasparri sulla stampa e tanta distrazione su quella che è la prerogativa maggiore del suo incarico. Questa Agenzia gestisce il maggior sistema di istruzione nell'area mediorientale, con la presenza di almeno 700 scuole. Essa è il maggior fornitore di istruzione elementare,

dall'Agenzia con complicità e aperture all'antisemitismo che disonorano i funzionari che hanno collaborato a ciò. Mi piacerebbe, senza per questo chiamare in causa esplicitamente il nostro Governo, che ha facilitato la nomina del dottor Grandi, che ci fosse una maggiore attenzione da questo punto di vista. Questo è un punto importante della nostra mozione. Era inevitabile, d'altronde, che noi, in occasione di una visita di Berlusconi in Israele, richiamassimo quello che a nostro avviso è stato un grande merito dell'Italia: essersi opposta, in solitudine, insieme a Stati Uniti, Paesi Bassi, Slovacchia, Ungheria e Ucraina, al «Rapporto Goldstone». Non voglio infierire sulla persona del giudice Richard Goldstone. Si è saputo oggi che è un fervente dottrinario della pena di morte, che ha comminato con molto godimento nel suo Paese di origine. Gli attacchi personali ci sono del tutto estranei. Ma è triste che le Nazioni Unite abbiano, per l'ennesima volta, consentito che sotto la propria sigla si potesse, da parte di un'autorità non indipendente e sulla base di fatti rivelatisi falsi, rivolgere un premeditato atto di accusa e di condanna a senso unico allo Stato di Israele.

che nella nostra mozione ci sia uno spirito diverso da quello di una precedente politica italiana. Per noi le Nazioni Unite su questa materia non sono un buon punto di riferimento: non non certo perché sono una tribuna che ospita Ahmadinejad ogni anno - è suo diritto prendere la parola - ma perché evocano l'episodio più vergognoso della storia occidentale, quando nel 1975

e ci fu solo un grande democratico, l'ambasciatore Patrick Moynihan, ad esprimere il proprio dissenso. ricordo storico, antico, che però mi è parso evocato, almeno come sentimento, in molti dei punti in premessa della nostra mozione. *(Applausi

la nostra prima preoccupazione concerne il programma nucleare perseguito dal Governo iraniano. e le rivendicazioni iraniane circa l'arricchimento dell'uranio costituiscono uno dei principali motivi di allarme, specialmente se uniti alle gravi dichiarazioni che spesso si sentono dai principali esponenti del Governo iraniano, dichiarazioni antisemite e sicuramente

non deve essere confuso e nemmeno interpretato come ostilità e inimicizia nei confronti di altri Paesi, ma sia ben chiaro che non possono essere tollerate le minacce, né ammessi atteggiamenti

Il problema nei confronti dell'Iran nasce proprio in seguito a questi atteggiamenti quotidianamente aggressivi nei confronti di Israele. Ciò genera inevitabilmente un sospetto e un allarme: che il Governo iraniano possa usare quello che chiama programma di arricchimento dell'uranio per scopi offensivi nei confronti anche, e soprattutto, del popolo e del territorio israeliani. Israele invece, va ribadito - come del resto la Palestina - ha diritto non solo di essere riconosciuto, ma di poter vivere

Fa bene ricordare che le 47 delegazioni convenute a Washington per il *summit* sulla sicurezza nucleare, il 12 aprile scorso, hanno dato il loro sostegno al piano del Presidente americano per ridurre nel giro dei prossimi quattro anni i quantitativi di uranio altamente arricchito e di plutonio disseminati nel nostro pianeta, in modo da garantire che tali materiali non cadano nelle mani di Paesi che possono essere considerati ad alto rischio o, peggio ancora, nelle mani di gruppi di terroristi, giungendo così alla successiva firma del nuovo Trattato sulla riduzione delle armi nucleari, che ha preso il nome di Start 2*.*

va in direzione opposta a quanto siglato nel Trattato Start 2. Un altro punto focale della mozione riguarda il richiamare l'attenzione

questo Corpo, in cui si raggruppano i cosiddetti pasdaran, riveste ormai un ruolo di primo piano sia nel sistema politico - infatti i suoi affiliati all'interno delle varie amministrazioni e non solo locali - sia sul piano militare. Si ritiene che i pasdaran possono svolgere un ruolo volto ad acuire situazioni conflittuali nei territori mediorientali, ed anche questo è inevitabilmente fonte di grande preoccupazione internazionale. Anche per questo riteniamo necessario che si accresca la pressione diplomatica sul Governo di Teheran affinché accetti di aprire un negoziato con la comunità internazionale circa il suo programma nucleare. Un terzo punto, ripreso poi anche tra le richieste di impegno nei confronti del Governo, è che riteniamo che debba essere assolutamente respinta l'ambizione da parte dell'Iran di avere un posto nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

nonché considerate le recenti esecuzioni di cui sono state vittime un elevato numero di persone appartenenti alla minoranza curda residente in Iran. Infine, va ricordato che fino al 2013 l'Agenzia per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi verrà diretta proprio da un funzionario italiano, Filippo Grandi. questa dovrà essere l'occasione che ci può vedere protagonisti all'interno dell'Agenzia - istituita fin dal 1948 da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite - affinché essa contribuisca finalmente a facilitare anche un processo di pace in Medio Oriente tramite azioni evidentemente concrete, e dovrebbe dovrebbe essere l'occasione di far luce su alcune criticità - chiamiamole così - interne che quest'Agenzia ha manifestato in modo ormai chiaro.

questi diritti umani non li rispetta e li viola in continuazione; salvaguardare evidentemente la sicurezza e i diritti dello Stato di Israele,

e sostenere comunque l'attuale e la futura attività di Filippo Grandi, funzionario italiano alla guida dell'Agenzia

si corre il rischio che questa discussione così importante diventi un'occasione perduta

Sul primo punto, come tutti sappiamo, come il Governo italiano ben sa, siamo a un passaggio molto difficile e delicato: il processo di pace e i negoziati sono sostanzialmente bloccati e in questo quadro ciò che è stato considerato dalla comunità internazionale come la chiave di volta per la soluzione del conflitto, cioè la parola d'ordine «due popoli, due Stati», rischia di entrare pesantemente in crisi. Stanno venendo meno quelle risorse di fiducia che sono alla base di una possibilità di dialogo e di convivenza, ed è evidente per tutti che il tempo non lavora per una soluzione positiva.

resistenze e forze che vengono da parti diverse. La prospettiva della pace trova oggi delle resistenze che vengono sia da un'ala del Governo israeliano che si muove in un'altra direzione (ancora ieri il ministro degli esteri israeliano Lieberman dichiarava essere la Siria di nuovo un Paese dell'Asse del male, proprio mentre la comunità internazionale si muove per coinvolgere la Siria in un nuovo negoziato)

Stati». Dobbiamo sapere se siamo in grado di muoverci con determinazione per contrastare queste tendenze e favorire quelle forze che si muovono invece nella direzione di un negoziato.

un elemento di raccordo come capitale storica delle diverse religioni e sul fatto che il suo destino non sia segnato con atti unilaterali. Allo stesso modo, mi pare che la comunità internazionale si stia muovendo per favorire un accordo che dia ai ai palestinesi la possibilità di una rappresentanza unitaria, che, chiudendo e risolvendo la contraddizione che da troppo tempo attraversa quel mondo, permetta alla comunità internazionale e allo stesso Governo israeliano di avere interlocutori attendibili in un negoziato.

e oggi c'è bisogno di una comunità internazionale che si muova in questa direzione e che aiuti il lavoro delle sue stesse istituzioni, a partire dalle Nazioni Unite.

ricordo che un funzionario italiano alle Nazioni Unite è un funzionario delle Nazioni Unite: non c'è nessuna guida italiana dell'UNRWA, c'è una guida delle Nazioni Unite che, per fortuna, è attribuita ad un dirigente italiano. A noi questo sembra il punto fondamentale

in forme inaccettabili, e soprattutto - lo voglio sottolineare, signor sottosegretario Mantica - in violazione di quei trattati internazionali, come la Convenzione sui diritti civili e politici, che lo stesso Iran ha sottoscritto. Non spetta a noi decidere quale sia la Costituzione iraniana, quale il rapporto tra politica e religione da loro stabilito, ma spetta a noi chiedere che i trattati che sono stati sottoscritti, gli impegni internazionali che sono stati firmati vengano rispettati. signor sottosegretario Mantica, credo che ci sia un problema per il Governo italiano come per la comunità internazionale: quello di chiedere che nell'agenda del confronto con l'Iran non trovi spazio solo la questione del nucleare, come fino ad oggi è stato, ma che anche quella dei diritti umani e delle libertà libertà acquisti un suo spazio e un suo ruolo. Naturalmente - questo è il punto determinante - dobbiamo sapere a chi ci rivolgiamo, cari colleghi: quali sono i nostri punti di riferimento? Sono o no quelle forze che si stanno battendo per la democrazia, sapendo che sono forze complesse, che non sono uguali a noi, non hanno la nostra stessa visione della democrazia? Ci sono forze religiose, ci sono forze invece espressione di una società che chiede maggiore libertà, ci sono parti stesse dell'*establishment*, perché sia Karrubi che Moussavi, i leader di questa protesta, sono stati uomini dell'*establishment*. Ma se si vogliono sostenere quelle persone

tale orientamento nella mozione che il senatore Compagna ha testé illustrato; non trovo una parola che riconosca e che cerchi di capire come si possono aiutare le persone che si stanno battendo per la democrazia. La democrazia in Iran non verrà infatti dal di fuori ma, se verrà, partirà da un'iniziativa che riguarderà gli iraniani, le loro scelte e lo sviluppo delle loro possibilità. Possiamo fare molte cose:

è bene che questa discussione sull'Iran sia inserita nel quadro generale di una discussione sul disarmo, e noi chiediamo - lo diciamo nella nostra mozione e ci interesserebbe conoscere in merito il parere della maggioranza e del Governo

di rispettare il Trattato di non proliferazione, facciamo finta di non vedere che esistono potenze nucleari nella regione, come il Pakistan, l'India e la stessa Israele, che devono conformarsi ad un diritto internazionale per la formazione di regole che sole possono assicurare un quadro di iniziativa

dell'azione della comunità internazionale. Sono queste le questioni fondamentali sulle quali a noi pare che il Governo e il Parlamento, attraverso le sue prese di posizione, possano esercitare un ruolo, ed è su questo che aspettiamo dal Governo delle risposte.

l'Italia dei Valori ha voluto rappresentare, in breve, un quadro della situazione mediorientale, concentrando la nostra illustrazione su due punti focali, senza la pacificazione dei quali è impossibile immaginare un futuro di pace a medio termine per tutta l'area: parlo dell'Iran e della zona israelo-palestinese. Vi enucleo alcuni punti della mozione. Il 10 maggio 2010 l'Organizzazione per la liberazione della Palestina ha approvato i cosiddetti colloqui indiretti con Israele, aprendo la strada ad un negoziato vero e proprio, che dovrebbe svolgersi nei prossimi quattro mesi, ridando slancio alla mediazione di pace americana portata avanti dall'inviato americano in Medio Oriente George Mitchell. Il negoziato che si sta avviando in questi giorni per il tramite dei colloqui indiretti - che si propone di superare l'interruzione dei colloqui diretti dovuta agli insediamenti israeliani nei territori dove i palestinesi intendono dar vita a un loro Stato, nonché all'annuncio di Israele del programma per costruire nuove case a Gerusalemme Est, altra area pretesa dai palestinesi - dovrebbe riguardare tutte le questioni relative allo *status* finale dello Stato palestinese, tra le quali la demarcazione delle frontiere, così come le garanzie di sicurezza per Israele. Durante la visita in Siria del presidente russo Medvedev, svoltasi solo due giorni addietro a Damasco, la Federazione Russa si è impegnata a riportare il processo di pace arabo-israeliano «sulla base legale internazionale vigente», con l'obiettivo di arrivare alla creazione di uno Stato palestinese indipendente, che possa esistere pacificamente a fianco di Israele. L'impegno ha registrato la disponibilità della Siria a compromessi in nome della pace, ma «ad eccezione dei casi che vanno a detrimento della sovranità di una o dell'altra parte». A quasi un anno dal famoso discorso del presidente statunitense Obama al Cairo, che tante attese aveva suscitato nella comunità internazionale e in particolare nel mondo arabo, occorre segnalare gli scarsi risultati raggiunti e la permanente incertezza sul futuro della pace in Medio Oriente, riconosciuti dallo stesso Obama, che ha ammesso che la situazione si è rivelata più complicata del previsto. Tuttavia, nonostante le palesi diffidenze del Governo statunitense nei confronti di quello israeliano, Obama grazie anche alla mediazione del ministro della difesa israeliano Barak, in luogo del più ostile ministro degli esteri Lieberman - ha trovato l'accordo per un congelamento di fatto di nuovi importanti progetti nella parte araba araba di Gerusalemme, almeno per i quattro mesi dei negoziati indiretti, anche se pubblicamente i leader israeliani continuano ad affermare il contrario, ed al contempo ha promosso altre misure di *confidence building* verso i palestinesi, quali il rilascio di prigionieri e la ulteriore rimozione di blocchi stradali. Per quello che riguarda le speranze, dobbiamo dire che gli Stati Uniti - ripartendo dalla «politica dei piccoli passi», con l'auspicio che questa possa riavvicinare palestinesi ed israeliani incoraggiandoli ai sopracitati negoziati - si stanno adoperando per ripresentare un piano di pace che, con l'appoggio della Federazione Russa, dell'Unione europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, riesumi i «parametri di Clinton» presentati a Camp David nel 2000 e rispolveri il vecchio negoziato tra Abu Mazen e Olmert del 2008. Tuttavia, la situazione politica interna dei due popoli in contesa non è certo delle più facili nell'ultimo cinquantennio. L'instabilità e l'incertezza palestinese, dovute principalmente alla frattura ancora non ricomposta tra Fatah e Hamas, frattura strumentalizzata da più Stati esteri tramite l'appoggio all'una o all'altra parte, rappresentano indubitabilmente un grosso limite al buon esito di un negoziato, purtroppo spesso portato avanti da interlocutori che, nel migliore dei casi, non rappresentano più della metà del popolo palestinese. Allo stesso modo i forti contrasti degli ultimi mesi tra gli Stati Uniti ed il Governo Netanyahu, dovuti principalmente alla politica radicale di non celata intransigenza nei confronti dei palestinesi, impersonata dalle posizioni oltranziste del ministro degli esteri Lieberman, non permettono di ritenere che il Governo israeliano possa gradire un piano di pace di tale portata, senza mettere in discussione la sua stessa tenuta. È oggettivamente imprescindibile, ai fini della riuscita del negoziato, l'appoggio di tutti i Paesi limitrofi ai contendenti e, quindi, la necessità di creare un quadro regionale stabile e ben disposto al negoziato.

La situazione è innegabilmente molto complessa e, rispetto a solo 10 anni fa, colleghi, possiamo dire che le speranze si sono affievolite, e purtroppo anche l'impegno della comunità internazionale rispetto al 1990 è sceso:

Un altro fattore di grande instabilità, a tutti i livelli, in Medio Oriente è rappresentato dall'Iran, grande potenza regionale islamica, sconvolta al proprio interno dalle recenti proteste seguite alla rielezione, contestata, di Ahmadinejad, soffocate nel sangue dall'*ayatollah* Khamenei, che si è rifiutato di annullare il risultato delle elezioni, ed hanno acuito ancora di più la crisi tra l'Iran e la comunità internazionale, accusata da Ahmadinejad di sostenere e foraggiare i contestatori. La politica della mano tesa inizialmente proposta dagli Stati Uniti ha incontrato l'ostracismo di un regime delegittimato dalla sua stessa opinione pubblica, che non può permettersi concessioni o trattative di tipo democratico, ma che al contempo cerca in tutti modi di creare o consolidare contatti con importanti attori della comunità internazionale, al fine di poter proseguire nel suo programma di indipendenza energetica, sviluppo militare ed aerospaziale. Cari colleghi, molto probabilmente, sino a quando la Repubblica islamica non ufficializzerà la sua posizione, i membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, con l'aggiunta della Germania, continueranno le consultazioni sulle eventuali sanzioni, i cui esiti sono incerti. Non possiamo dimenticare, infine, che ogni giorno in Iran vengono violati importanti ed elementari diritti umani. Per questo, come Italia dei Valori impegniamo il Governo ad essere in sede europea attivo ed efficace protagonista, al fine di ottenere che l'Unione europea, senza defezioni e tentennamenti di singoli Stati membri e senza passivo attendismo, collabori fattivamente con gli Stati Uniti nella difficile ripresa del processo di pace in Medio Oriente, mettendo in gioco tutte le proprie risorse, in termini di rapporti diplomatici ed economici, nei confronti dello Stato di Israele, dei palestinesi e degli Stati confinanti, non mancando di censurare la politica di quegli Stati che si ostinano a non voler riconoscere l'esistenza dello Stato di Israele. Ogni sforzo, per la soluzione del conflitto in Medio Oriente, è fondamentale non solo per la loro pace e sicurezza, ma anche per la nostra.

onorevoli colleghi, innanzi tutto ringrazio il senatore Compagna che ha giustamente lamentato, con la consueta

estera. Onorevoli colleghi della maggioranza, non vi è dubbio che nel vostro documento vi siano punti assolutamente condivisibili, forse più

facendo in modo di svincolare tale tema dalle questioni di politica interna. È chiaro a tutti che negli ultimi anni il rapporto con Israele è stato spesso utilizzato come una sorta di cartina di tornasole per dimostrare un certo affiancamento dal punto di vista democratico. In realtà, non vi è alcun bisogno di legittimare la destra di questo Paese, che noi riteniamo e speriamo sia una destra conservatrice europea, al pari dei gollisti e dei conservatori britannici nati dalla lotta al nazismo e al fascismo; dunque, non credo vi sia più bisogno di questo tipo di vicinanza. Dovremmo invece analizzare il tema di Israele e della Palestina come un tema oggettivo di politica estera,

la pace prima che il loro Stato-Nazione, l'Italia può dare su questi temi una svolta al proprio impegno, soprattutto prescindendo dalle questioni di politica interna. Questo è l'unico modo per poter trovare un'intesa su un documento comune.

Vorrei però soffermarmi sul cosiddetto processo di pace in Medio Oriente. All'indomani della prima Intifada, i radicali organizzarono un consiglio generale del loro partito a Gerusalemme, pubblicando su tutti i maggiori quotidiani israeliani un appello affinché Israele divenisse pienamente uno degli Stati membri dell'allora Comunità europea. una proposta che noi radicali non abbiamo mai cessato d'avanzare, poiché si riteneva allora - e riteniamo ancora oggi - che, nell'affermazione dei principi che hanno fondato l'Unione europea, vi possa essere la speranza della promozione della pace, della giustizia giusta ed equa e del progresso umano. Alle guerre e ai conflitti, anche di ispirazione o giustificazione religiosa, occorre rispondere con politiche basate sui principi fondativi della comunità internazionale, quelli della Dichiarazione universale dei diritti umani e di tutti gli altri documenti che negli ultimi sessant'anni ci hanno fatto acquisire la nozione dell'inviolabilità delle libertà individuali. Su questa analisi Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, dal loro confino dell'isola mediterranea di Ventotene, elaborarono quel Manifesto che chiedeva con forza la creazione degli Stati Uniti d'Europa per prevenire un'altra guerra atroce, senza necessariamente dover aderire ad uno dei due schieramenti che, in quegli anni, stavano combattendo il nazi-fascismo. Con quel documento quei radicali *ante litteram* andavano però oltre: individuavano nella sovranità assoluta degli Stati il problema e non la soluzione contro persecuzioni ed oppressioni. Nel 2010, oltre che nella nostra Europa, l'obiettivo del depotenziamento del potere distruttivo della sovranità nazionale resta di pressante attualità. Nella sua visita in Israele nel febbraio scorso, più volte ricordata questa mattina, il presidente Berlusconi ha definito un sogno vedere un giorno Israele nell'Unione europea. Perché non si rintraccia niente di tutto ciò nella mozione della maggioranza? A leggere gli impegni che si chiedono al Governo, pare quasi che i problemi principali ed esclusivi di Israele siano da una parte la minaccia dell'Iran e dall'altra le attività mascherate dell'agenzia dell'ONU UNRWA. Posto che è sempre utile ed opportuno amministrare in modo efficace e trasparente i soldi dei nostri contribuenti (quindi i soldi pubblici), ci vuole uno scatto della politica per affrontare la questione alla radice e corrispondere alle richieste dei popoli di quella parte del mondo. In più occasioni, negli ultimi cinque anni, sondaggi della Commissione europea (che non può essere sicuramente tacciata di filosionismo) e della Fondazione Konrad Adenauer hanno fatto emergere una realtà che vede gli israeliani desiderosi di diventare cittadini europei. Una buona metà di loro già lo è in virtù della provenienza famigliare o delle parentele: oggi vorrebbero divenirlo in virtù del loro essere israeliani. Per rendere un servizio alla ricerca della pace tra israeliani e palestinesi, ma anche per i siriani, i libanesi, i giordani e gli egiziani, occorre dar loro la possibilità di dibattere di questa richiesta, di approfondire e condividere con l'opinione pubblica euro-mediterranea la prospettiva di spostare i confini dell'Unione europea dall'Oceano Atlantico al Mar Morto, dal Mare del Nord al Mar Rosso. Non si tratta quindi di prendere una parte piuttosto che l'altra, né di volersi ergere al ruolo di mediatori: si tratta di chiedere l'affermazione del diritto internazionale per i presunti

le aspirazioni di milioni di azeri, kurdi, arabi, ahwazi, baluci, turcomanni e assiri, di cui non dobbiamo mai dimenticarci, poiché negli ultimi anni stanno sviluppando politicamente la loro opposizione al Governo. Per questo la delegazione radicale - in particolare, il senatore Perduca sta lavorando al riguardo - li ospiterà per un dibattito

forse, iniziare a utilizzare come parole chiave per affrontare proprio alla radice la questione «Israele nell'Unione europea» farebbe compiere un passo avanti al dibattito.

rispetto alla situazione mediorientale e a come immaginare di proseguire il processo di pace.

però non possiamo che assumere la situazione attuale (partendo dalle iniziative dell'ONU, degli Stati Uniti, del Quartetto, dell'Unione europea), inserirci in questo filone e dare una mano perché le cose possano ricominciare a procedere.

ed è da questa mattina che cerco di capire come riuscire a fare una sintesi di queste venti pagine di documenti che sono state scritte. Poi entrerò nel merito delle osservazioni, ma consentitemi di inquadrare il problema, dicendo che, ancora una volta, si ripresenta un metodo molto italiano di ragionare di politica estera, che potrei riassumere in questa definizione. La politica estera italiana ha una caratteristica: non è estera, ma è una politica che risente molto di quelle che sono le legittime posizioni dei Gruppi parlamentari. Lo si legge soprattutto se si osserva il rapporto con il presidente Obama. Io, che sono sempre stato filoamericano, fin da bambino, sono molto imbarazzato di questo amore verso gli

Quanto fa il Presidente degli Stati Uniti è un atto responsabile del Governo degli Stati Uniti. Noi, come Paese, dobbiamo osservarne le conseguenze nel nostro interesse, nel quadro di questa alleanza storica che certamente nessuna delle parti, in questa Assemblea, vuole venga

gli impegni finali non sono così diversi da poter dire sì e no in maniera *tranchant* su una mozione piuttosto che su un'altra.

avvertito da tempo l'esigenza di cambiare l'immagine dell'Agenzia e del suo modo di agire sostenendo noi, sostenendo noi, che siamo tra coloro che danno un contributo a detta Agenzia, che questa figura di assistenzialismo puro alla popolazione rifugiata palestinese, che pure è un'opera meritoria, non è sufficiente.

Questo, secondo noi, è il grave difetto dell'UNRWA, che in maniera, osiamo dirlo, molto passiva per molti anni ha incassato i contributi ed ha erogato servizi di assistenza, perdendo nel tempo il significato ed il ruolo politico per cui era nata.

Non voglio entrare nella polemica, né esprimere opinioni personali su quanto è avvenuto durante l'operazione a Gaza ma, senza entrare in quel dibattito, voglio dire che come cittadino italiano e membro di questo Governo sarei lieto un giorno di vedere un libro di scuola delle elementari di un bambino palestinese che riportasse la presenza di Israele nel territorio geografico.

vicino. Altrimenti, se non si insegna che esiste anche Israele, il bambino stesso crescerà pensando che quegli altri, diversi, che sono lì, non appartengono a quel territorio e alla sua storia.

che nel dibattito che avviene nelle sedi ONU di Ginevra il problema del mondo sia sostanzialmente Israele. È perlomeno anomalo, nel senso che secondo noi qualche altro problemino nel mondo vagamente esiste. Ma pare che a Ginevra Israele sia considerato il responsabile di tutto

il fatto di aumentare il numero dei partecipanti e quindi di includere è un moto necessario. Infatti, dobbiamo far entrare in questa comunità il maggior numero possibile di Stati membri e di popolazioni perché, da un certo punto di vista, ciò significa che il nostro modo di ragionare diventa un elemento di dialogo da altre parti, ma talvolta questa inclusività porta a posizioni che non possono essere condivise.

è più bravo il Ministro della difesa piuttosto che il Ministro degli affari esteri. Siamo di fronte ad un Governo israeliano che ha mutato atteggiamento rispetto al precedente in una logica anche comprensibile dal punto di vista politico, visto che la maggioranza è passata da Kadima ad un'altra formazione politica, che ha sempre detto esattamente cosa pensa. Peraltro non dobbiamo nemmeno, in questo nostro dibattito, dimenticare che Israele è l'unica democrazia vera del Medio Oriente, dove i Governi sono l'espressione legittima di una volontà popolare che si manifesta secondo gli standard europei.

dobbiamo operare, sapendo che da una parte c'è un Governo israeliano molto rigido, ma dall'altro non c'è nessun cambiamento, nemmeno da parte di quelle strutture che hanno certamente un significato politico. Mi riferisco ad Hamas e ad Hezbollah, che non si capirebbe cosa sono se non si sapesse che sono anche l'espressione di una parte politica, ma che hanno al loro interno una struttura tipicamente militare e terroristica, perché nel fare politica ritengono che il terrorismo sia uno strumento di dibattito e di confronto politico. In questo viene la condanna.

che è Paese che pretendo di conoscere abbastanza bene e che ho sempre considerato una grande potenza regionale, che deve svolgere un grande dialogo all'interno del dibattito sul Medio Oriente, ma che non vuole evidentemente immaginare di essere un interlocutore affidabile - come spero diventi al più presto se continua in una azione di ponte e di sostegno nei confronti di due formazioni che non sono solo politiche ma anche terroristiche. Se ciò che ha affermato il Governo in questo momento grosso modo riprende i temi che si sono espressi nel dibattito e nella lettura dei documenti, mi sento di rivolgere - consentitemi - da collega del Senato un appello ai miei colleghi. Credo che quest'Aula abbia una grande tradizione da difendere anche a livello di comportamento:

ad una votazione delle quattro mozioni. E vi dico onestamente che il Governo sarebbe seriamente imbarazzato a rispondere alla domanda, corretta, del Presidente di esprimere il parere sulle mozioni,

dare un'indicazione seria e importante di impegno del Governo italiano su materie certamente delicate, credo che il Senato nel suo complesso farebbe un

apprezza. Ovviamente il dibattito sulla nostra mozione - voglio ringraziare il senatore Compagna per il suo intervento e il senatore Malan, che si accingeva a fare una dichiarazione di voto che evidentemente non avrà luogo in questa fase

essa era incentrata su alcune questioni: il comportamento del regime iraniano; il comportamento di alcuni movimenti (Guardiani della rivoluzione ed altri) all'interno dell'Iran; il collegamento di tesi fondamentaliste e di intolleranza con gruppi come Hezbollah e poi Hamas in altri contesti; le polemiche che hanno investito anche il comportamento di alcune Organizzazioni internazionali. Noi presentammo la mozione diverso tempo fa: non c'è dubbio che ulteriori fatti si sono aggiunti, e quindi le altre mozioni hanno fotografato anche un aggiornamento della dinamica degli eventi. Il nostro intento - lo sottolineo nell'accogliere l'invito

un rinvio a data da destinarsi: ma questo è un problema del Senato, e non del Governo. Quindi, auspichiamo che la Presidenza possa assicurarci una rapida calendarizzazione. Prendiamo comunque atto che su alcuni temi, sul fondamentalismo come minaccia al Medio Oriente e sul comportamento del regime iraniano, con le minacce che Ahmadinejad e l'Iran rivolgono in continuazione soprattutto nei confronti dello Stato di Israele, ci sia necessità di un'azione internazionale pressante, decisa, non minimalista, di cui l'Italia si è già fatta protagonista in varie occasioni. Essa riguarda sia i diritti della popolazione iraniana - abbiamo visto tutti le immagini di quello che sta avvenendo - sia le preoccupazioni,

Signor Presidente, noi accogliamo con favore e, mi consenta di dirlo, anche con un certo sollievo la proposta del sottosegretario Mantica. Dico sollievo perché oggi ci saremmo trovati nella situazione di non poter votare la mozione della maggioranza, non tanto per lo spirito, che comprendiamo e anche apprezziamo, in alcuni passaggi, ma per la sua formulazione tecnica, a nostro avviso bisognosa di un approfondimento e di una una migliore attenzione. Del resto (è stato detto anche dal senatore Compagna e ripetuto adesso dal presidente Gasparri) si tratta di una mozione che era nata in un determinato contesto, e oggi ci troviamo in un contesto parzialmente diverso. Tuttavia, non avremmo voluto votare contro, non avremmo voluto dividere il Parlamento, in particolare il Senato italiano, su due grandi questioni, forse le due principali di politica internazionale in questo momento,

Siamo un grande Paese, ma anche una media potenza: non possiamo illuderci di essere risolutivi in nessuna di queste due grandi questioni. Abbiamo però un ruolo che possiamo svolgere nella linea di fondo tradizionale di politica estera del nostro Paese,

recuperi una capacità di protagonismo, una capacità più assertiva, e sappiamo quanto siamo lontani da tale obiettivo. Nonostante il Trattato di Lisbona abbia introdotto la figura del del responsabile della politica estera, vediamo ancora quanta strada ci sia da fare perché l'Europa possa, come tale, esprimere una posizione forte. Il secondo grande pilastro è l'amicizia, la solidarietà transatlantica con gli Stati Uniti d'America. Anche questa è una costante della politica estera italiana che scavalca sia i Governi italiani che le Amministrazioni americane. caposaldo è il multilateralismo, e quindi il nostro pieno sostegno alle organizzazioni delle Nazioni Unite come grande luogo di incontro tra i popoli, per la costruzione di un assetto fondato sul diritto e non solo sulla forza nei rapporti internazionali. Naturalmente nessuno di questi tre pilastri significa un'adesione acritica. È evidente che si può e si deve discutere di come l'Europa concretamente agisce di di fronte a tali problemi; si può e si deve discutere di come le amministrazioni americane si comportano, ed anche di come le Nazioni Unite concretamente agiscono, direttamente o attraverso le loro Agenzie: nulla è precluso ad una discussione approfondita e seria. Credo però che questo debba essere lo spirito che ci guida, e allora penso che arrivare oggi ad un voto diviso in quest'Aula sarebbe stato

in Commissione, per arrivare possibilmente ad un testo unitario, o comunque a dei testi più maturi, che possano consentire al nostro dibattito di instradarsi verso una posizione costruttiva che possa dare al Governo

testo, ad un testo condiviso, proprio per imprimere la necessaria e opportuna forza affinché da questa Aula arrivi un messaggio a livello internazionale, non solo serio, ma sempre più importante e sempre più pieno di positività per un'area che evidentemente sta soffrendo una crisi che da troppo tempo incombe.

duro, forte, chiaro e netto a un nucleare militare, anche e soprattutto se se in uno Stato come quello iraniano che in questo momento lancia messaggi non proprio pacifici nei confronti di altri Paesi, in modo particolare nei confronti

Invece, un sì importante e forte, anch'esso chiaro, al diritto di Israele, come anche del popolo palestinese, di vivere non solo dignitosamente

*(IdV)*. Signor Presidente, anche l'Italia dei Valori accetta l'invito del Governo. Lo accogliamo, come Italia dei Valori, per rinviare il dibattito per un approfondimento che risulta necessario e puntuale. Credo sia giusta la considerazione del Governo

E poiché avremmo deciso di votare a favore di tutte e quattro le mozioni, perché i dispositivi erano sicuramente condivisibili, e avremmo considerato

che le indagini successive delle procure di Firenze e di Perugia hanno messo in luce. Già il 5 marzo, signor Presidente, onorevoli colleghi, ponevo dubbi sugli appalti, perché i lavori sono stati aggiudicati previa gara esperita dal commissario delegato alle opere pubbliche e private per i mondiali di nuoto, ingegner Claudio Rinaldi, subentrato all'ingegner Angelo Balducci, ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ponevo quindi tutta una serie di questioni riguardo alla mancanza di trasparenza da parte anche della Protezione civile. In particolare, citavo una sentenza della Corte costituzionale, la n. 127 del 1995, che afferma che il potere di deroga alla normativa primaria

un senso di giusta distanza dalla commistione che emerge. Concludo, signor Presidente, citando alcuni giornali di oggi: